nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

maggioranza coinvolge quasi interamente le forze del Parlamento, di avere la possibilità di fare un'opposizione organizzata, anche attraverso le forme indicate dal Regolamento,

o, peggio, il diniego alla costituzione di questa componente comprime la possibilità di fare opposizione in forma organizzata, non come singoli, ma come collettivo, in rappresentanza di una collettività maggiore presente nel Paese e che non è rappresentata in

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha terminato i suoi lavori poco fa senza conferire il mandato al relatore. Eravamo informati, fin da ieri, che probabilmente il Governo avrebbe

senza le quali si rischiava di rimanere esclusi dalla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Ciò evidentemente sarebbe stato un colpo per tutto il nostro sistema sportivo e per il nostro sistema Nazione, per tutti coloro che nello sport vedono un modo per migliorare la propria condizione di vita, la propria salute e il proprio spirito, ma anche per tutti coloro che, da appassionati, in questo periodo di difficoltà così elevata, hanno trovato nello sport uno sfogo, uno sbocco e una possibilità di evadere da una quotidianità che evidentemente è molto difficile.

il secondo redistribuisce le risorse tra CONI e la società Sport e salute SpA; il terzo indica la clausola di neutralità finanziaria e il quarto disciplina i tempi di entrata in vigore del suddetto decreto.

in sede di conversione, ma probabilmente anche necessario, perché, non avendo più molto tempo, potremmo rimpiangere il fatto di non avere iniziato subito a discutere di ciò che sarebbe necessario per il nostro sistema sportivo. Ho detto prima che lo spunto era stato la partecipazione ai giochi olimpici e, secondo me, questo mi consente di fare già un primo collegamento tra l'importanza dello sport e la quotidianità di tutti noi.

ma può essere praticato da tanti appassionati che, così facendo, migliorano non solo il proprio stato psichico, ma anche le proprie condizioni fisiche. È universalmente riconosciuto, infatti, che lo sport sia probabilmente il più antico, il più efficace e il più salutare metodo di vita. Lo definisco "metodo" perché è dimostrato che chi fa regolarmente attività sportiva ne trae giovamento e e arriva a migliorare anche le proprie condizioni fisiche. Tutto questo per dire che il decreto-legge al nostro esame, che non poteva che essere strutturato in maniera così semplice, essendo finalizzato al soddisfacimento di un'esigenza specifica,

amatoriale o seguono lo sport pur non praticandolo e soprattutto quanto lo sport può essere importante per il nostro spirito di corpo, per la capacità di aggregazione che crea

per le vittorie che riporta, ecco che ci sentiamo orgogliosi e fieri del fatto che rappresenti la nostra stessa Nazione. Da marchigiano potrei fare un altro esempio: pochissime persone seguono il *volley*, ma, nel momento in cui la Lube ha ottenuto certi risultati a livello internazionale, tutti ci siamo sentiti orgogliosi di avere una simile realtà nel nostro territorio. Tutto questo per dire che lo sport

solo la qualità della nostra vita, ma anche le relazioni sociali e i nostri rapporti con gli altri, e quindi far sì che si possa uscire meglio, più rapidamente e non dico in maniera indolore - perché temo che potrebbe non essere possibile - ma in maniera più agevole, sì, dalle difficoltà che stiamo vivendo. Considerando il poco tempo che ho a disposizione, mi permetto di indicare alcuni spunti di riflessione che, secondo me, dovrebbero essere contenuti in un provvedimento successivo a questo che ci troviamo a discutere oggi, che, per evidenti motivi, non avrebbe potuto contenere Penso alle 19 discipline sportive associate, che strutturalmente e funzionalmente sono come federazioni, ma non hanno tale rango. Questo

qualifica, non hanno la possibilità di attingere a determinati fondi. Sia chiaro, però, che ciò che propongo non è di consentire anche a queste discipline

anche a livello internazionale, si è accettato di avviare sperimentazioni per far sì che alcune possano partecipare alle Olimpiadi; hanno centinaia di migliaia di iscritti in tutta Italia

dovrebbe impegnare maggiori risorse anche per il soddisfacimento delle loro necessità, al fine di consentire a tutti coloro che si vedono rappresentati in queste discipline di praticare lo sport che amano, senza le limitazioni che adesso hanno. Un ulteriore vantaggio sarebbe

il tempo è troppo poco e non me lo consente. Spero che si rilevi lo spirito positivo di questo intervento, che vuol essere un incentivo affinché non si perda il tempo che non abbiamo per arrivare alla disciplina di un settore

Signor Presidente, devo purtroppo constatare come la materia dello sport sia trattata in modo a dir poco ambiguo dall'odierna maggioranza. Provo a ricostruire brevemente i fatti. Il decreto-legge n. 5 del 2021 è stato l'ultimo atto approvato dal Governo Conte-*bis* per evitare l'apposizione di sanzioni da parte del Comitato olimpico internazionale che avrebbero probabilmente comportato l'assenza della bandiera italiana ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo. Il contenuto dell'atto, tuttavia, avrebbe potuto essere ben diverso. Basti guardare il testo degli emendamenti,

Nessuna proposta parlamentare, però, è stata approvata, perché la Commissione ha deciso a maggioranza - ovviamente con noi contrari - di rimettere all'Assemblea, e quindi al voto di fiducia, il decreto così com'era. Chiedo quindi a me stessa, all'Assemblea e a tutti i cittadini interessati quale sia la ragione per cui il decreto aumenta inopinatamente il numero dei dirigenti del CONI, incrementando d'un tratto il rapporto tra funzionari e dirigenti: perché mai dare al Comitato maggiori risorse, sottraendo contributi pubblici a sport e salute,

Perché trasferire la proprietà di un bene immobile di particolare rilevanza come il centro sportivo "Giulio Onesti" di nuovo nelle mani del CONI? Ricordo come già la riforma dello sport voluta dall'ex ministro Spadafora sia rimasta totalmente monca, perché sul tema del rinnovo dei mandati del Presidente del CONI non è stata trovata una quadra. Per fortuna, è stato vanificato il rischio di un'immotivata retromarcia, che pure era stata paventata sugli altri decreti delegati approvati *in extremis.* L'emblema dell'unione promiscua delle nuove forze che sostengono il Governo Draghi può essere sintetizzato in questo accadimento: in Commissione istruzione,

dopo che l'atto governativo aveva spostato la competenza al Dipartimento per lo sport di Palazzo Chigi, ovvero di fatto ne chiedeva l'abolizione. Probabilmente, però, per mandare a segno quel pacchetto di riforme senza troppi intralci si è dovuto cedere qualcosa al CONI e lo si è fatto a stretto giro, nel decreto-legge n. 5 del 2021. Mi riferisco sia alla fase di stesura del testo del decreto-legge, sia alla fase di conversione, nella quale è stata preclusa ai senatori l'approvazione di modifiche che avrebbero riportato l'esito definitivo entro confini di maggiore imparzialità ed equità. Lo dico con rammarico, ma la posizione originaria del MoVimento 5 Stelle sulla *governance* sportiva non prevedeva davvero maggiori contributi pubblici e trasferimento delle proprietà di beni immobili al CONI, una dotazione di personale aggiuntiva rispetto a quella attuale e un aumento immotivato del numero dei dirigenti. Ricordo che, durante la scorsa legislatura, il tema del limite al numero dei mandati era dirimente. Si dichiarava di voler mantenere il limite inderogabile dei due mandati per i più importanti incarichi pubblici, dal parlamentare ai gradi apicali di enti o società pubbliche, CONI e federazioni sportive comprese, e si diceva che la riforma, che aumentava da due a tre i mandati dei vertici federali e del CONI, compreso il Presidente, non solo non avrebbe garantito la normale alternanza delle delle cariche presidenziali e dirigenziali nel mondo dello sport, bensì le avrebbe cristallizzate, come se lo sport fosse una questione privata, quasi personale, sulla quale i partiti sono interessati esclusivamente ad esercitare ai fini del consenso la loro influenza e il loro potere. Ebbene, noi parlamentari della componente "L'alternativa c'è" vogliamo rappresentare quella posizione che già era di un movimento che non c'è più e che una frase di quel programma originario, ormai del tutto disatteso, sintetizza bene: «liberare il mondo dello sport da interessi che nulla hanno a che fare con la crescita del sistema sportivo italiano, adoperandosi affinché i vertici delle più importanti amministrazioni vengano scelti secondo criteri meritocratici adeguati a garantirne il buon andamento». Le nostre proposte emendative infatti presentavano un chiaro connotato politico, che era quello di ridurre le elargizioni fatte al minimo indispensabile, senza ulteriori indulgenze non dovute. Per queste ragioni, voteremo contro la conversione in legge del provvedimento, che rappresenta una decisa retromarcia rispetto alla direzione intrapresa finora in materia di sport.

colleghi, signori membri del Governo, il decreto-legge che discutiamo quest'oggi e che il Parlamento sarà chiamato a convertire in legge è stato uno degli ultimi atti del precedente Governo. Ricordiamo tutti il clima e le modalità con le quali il provvedimento fu deliberato. C'era grande preoccupazione, visto il campanello d'allarme lanciato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, che aveva infatti denunciato il rischio che gli atleti italiani potessero andare alle Olimpiadi di Tokyo senza il nostro tricolore e l'inno nazionale. una sanzione che il Comitato olimpico internazionale (CIO) avrebbe potuto comminare al nostro Paese, se non avessimo garantito, come poi è avvenuto con l'approvazione del decreto, l'autonomia di un organismo importante quale il CONI: una situazione umiliante. Tutto ciò avrebbe avuto conseguenze nefaste dal punto di vista sportivo e devastanti dal punto di vista dell'immagine del nostro Paese; è un aspetto che assume ancora più rilevanza, se pensiamo al peso e a ciò che il nostro tricolore rappresenta in un Paese come il Giappone, ma in generale in una zona geografica come l'Oriente, nella quale il *made in Italy* è sicuramente un marchio riconosciuto e riconoscibile. Solo l'approvazione in Consiglio dei ministri di tale decreto-legge ha dunque evitato il peggio. Resta però l'amaro in bocca per come è stata gestita l'intera questione, per le condizioni nelle quali si è dovuto in tutta fretta scongiurare un pericolo che un Paese serio, quale è l'Italia, non dovrebbe correre in nessun modo.

La pandemia ha avuto un impatto fortissimo per il tessuto produttivo ed economico, ma ha indubbiamente una rilevanza e un'incidenza importanti nelle nostre vite dal punto di vista non solo economico, ma anche sociale. Lo sport, come il mondo dell'associazionismo, ha senz'altro subito un durissimo stop forzato, al quale il Covid ci ha tutti obbligati. Se i massimi campionati sportivi hanno avuto la possibilità di continuare il proprio percorso con tutte le precauzioni previste dal Comitato tecnico-scientifico, di contro lo sport amatoriale e non professionista non ha avuto le stesse possibilità. Questo ci ha forse resi ancora più consapevoli di quanto lo sport eserciti in modo netto una funzione importante per la nostra vita. Mi permetta, signor Presidente, di aprire qui una parentesi,

non solo è un danno importante alla qualità della vita delle persone, ma ci dovrebbe indurre anche ad interrogarci sui criteri che il Comitato tecnico-scientifico ha deciso e deliberato per far sì che ad alcuni livelli ci si possa organizzare e si possa ripartire e ad altri no. Vorrei evidenziare che il Politecnico di Milano ha recentemente diffuso uno studio scientifico con il quale pone alcune questioni che valgono per lo sport, come per la scuola e per tutti gli spazi chiusi, quali ad esempio la ristorazione. Non c'è soltanto il distanziamento sociale quale parametro per definire i criteri per poter limitare la diffusione del virus. Per calcolare l'indice di probabilità di un contagio in un ambiente *indoor* si deve moltiplicare il quadrato della densità degli utenti per il tempo di ricambio del volume d'aria. Ora, signor Presidente, si comprenderà che anche dentro uno spazio chiuso dove si pratica sport è facilmente calcolabile questo parametro e lo si può confrontare con quelli della scuola, della ristorazione e dell'impresa. Invito il Comitato tecnico-scientifico e il Governo, rivolgendomi agli esponenti oggi qui presenti,

in un quadro siffatto, il Governo è stato chiamato a un intervento adottato *in extremis*, muovendosi in una fase complessa per il mondo dello sport, dovuta anche a una riforma che nel 2018 aveva dato vita a una sperequazione tra le funzioni e le risorse attribuite, da una parte, alla nuova struttura Sport e Salute SpA e, dall'altra, a quelle lasciate a disposizione del Comitato olimpico nazionale italiano. Quest'ultimo aspetto lascia sicuramente qualche perplessità, viste le immutate competenze e funzioni che vengono lasciate a un ente come il CONI, il quale nel corso della sua storia ha svolto un ruolo indubbiamente importante. In questa sede possiamo dirci che proprio tale impianto e le condizioni date ci hanno portato a indebolire e a mettere in discussione l'autonomia del CONI. Lo stesso Comitato internazionale olimpico (CIO) ha rappresentato all'Italia una serie di doglianze sul ruolo, la missione, l'autorità e la responsabilità del CONI, assoggettato al rispetto dei requisiti minimi della carta olimpica. È stato eccepito che il personale del CONI non potesse essere assunto e controllato da un'entità esterna riconducibile alla Sport e Salute SpA, ma che dovesse avere una propria dotazione organica e una propria struttura amministrativa. Questo decreto-legge mira a raggiungere tale finalità, garantendo la piena operatività del CONI, nonché la sua autonomia e indipendenza. L'articolo 1, comma 1, dispone infatti che il CONI sia messo in condizioni di avere una propria dotazione organica, in modo da essere pienamente operativo rispetto alle funzioni assegnategli. Messo in sicurezza questo aspetto e scongiurata la possibilità che gli atleti dovessero rinunciare a una bandiera e a un inno italiani, arriviamo alla situazione attuale, che chiama un nuovo Governo a gestire le fasi che verranno. Nella composizione di quest'ultimo, la casella della delega allo sport non è ancora stata assegnata. Mi auguro che ciò avvenga quanto prima. Al netto di chi avrà la responsabilità di occuparsi di un settore fondamentale per la vita della nostra Repubblica, penso che la conversione del decreto in esame sia solo il primo atto di un processo di riforma che impegnerà il Governo nei prossimi mesi e che dovrà vedere il Parlamento sempre protagonista. Signor Presidente, l'attualità di quest'oggi non può esimermi dal fare

adeguata le proprie funzioni, allo stesso tempo non possiamo non chiedere allo sport di mettere gli atleti nella condizione di esercitare la propria passione e anche la propria professione a livelli agonistici in maniera adeguata e dignitosa. La vicenda di Laura Lugli, la pallavolista del Pordenone che ha denunciato di non essere stata messa nella condizione di vivere la propria maternità come una qualsiasi lavoratrice, credo sia grave. *(Applausi)*.

e facciano lo sforzo necessario per garantire anche alle lavoratrici e alle professioniste di questo mondo così importante di svolgere la propria passione e la propria funzione con dignità, in maniera adeguata e nel pieno rispetto delle norme del nostro Paese, della nostra Costituzione e in maniera conforme e coerente con quello che le altre donne impegnate in altre professioni possono fare. siamo l'Italia e abbiamo l'obbligo di costruire un sistema che a tutti i livelli, nell'autonomia dello sport e nella dignità per chi svolge la professione sportiva ai massimi livelli, esiga di poterlo fare

quando è stata approvata la legge delega e si è consumato lo scontro, che è ancora

Parliamo di una rappresentazione sociale che investe l'attenzione di milioni di italiani italiani e di un settore - forse uno dei pochi del nostro Paese - ancora in grado di produrre grandi numeri di partecipazione. tale settore è stato spesso sottovalutato e nella nuova configurazione del Governo viene addirittura ignorato, con l'impossibilità di poter rappresentare le proprie esigenze e istanze e avere un

Noi di Fratelli d'Italia abbiamo subito sottolineato e denunciato che l'assenza di un Ministro dello sport come abbiamo verificato successivamente, addirittura la mancanza del conferimento di una delega in materia di politiche dello sport rappresentano un gravissimo *vulnus* del nuovo Governo. abbiamo subito anche una gravissima mortificazione in Commissione in quanto l'approvazione dei decreti legislativi senza il parere, seppur consultivo, della Commissione ha rappresentato un primo schiaffo.

che riguardano le materie di sua competenza sulle quali dovrebbe essere più facile trovare delle intese nell'interesse dei mondi che rappresentiamo, seppur nella legittima e sacrosanta diversità di visione culturale di cui ognuno di noi

Siamo al terzo provvedimento che arriva in Senato e il Governo Draghi si avvia già a consumare un *record*: due fiducie su tre provvedimenti. la dice lunga sul pensiero unico che vuole dominare questa fase che vive la nostra Nazione, con un partito, Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione, che tuttavia si sforza quotidianamente di fare proposte e portare avanti un'opposizione patriottica. Ma, anche al cospetto del nostro atteggiamento propositivo, ci viene letteralmente vietato di dare il nostro contributo. Riteniamo scandaloso che oggi si consumi in poche ore un voto di fiducia su questo provvedimento e che l'Assemblea non continui a lavorare nel pomeriggio e nella giornata di domani.

le manifestazioni che si stanno consumando fuori dai Palazzi ci danno una rappresentazione drammaticamente triste di quanto sta vivendo questo mondo, un mondo che ha come suo fatturato la passione e che è stato abbandonato a se stesso da un Governo che evidentemente non ha una visione univoca, un Governo che non ascolta le istanze. Ieri alla Camera il nostro partito ha presentato un emendamento

è stato respinto, ma sarebbe passato se chi si è sempre detto favorevole a questa soluzione non si fosse astenuto; vi assumete una grande responsabilità rispetto a un mondo che è stato lasciato solo e che non ha ricevuto indennizzi significativi. Si continua a dire "domani vedremo, non potete lavorare e domani vedremo". Rispetto a questo, vi diciamo con grande chiarezza che Fratelli d'Italia ci sarà sempre quando le decisioni saranno a favore

Signor Presidente, membri del Governo, grazie per essere qui. È già stato detto abbastanza su questo decreto-legge che oggi arriva in Aula. È stato detto soprattutto perché è arrivato in questo modo e cosa ci troviamo a votare oggi. Il Partito Democratico da sempre, votando contro la riforma Giorgetti, aveva detto che il nuovo sistema della società Sport e Salute SpA e del CONI, svuotato praticamente delle proprie prerogative, non ci convinceva e non era il modo giusto per affrontare il mondo dello sport e tutto il sistema educativo che sta al suo il Partito Democratico ritiene fondamentale. Dispiace quindi che si arrivi a convertire il decreto-legge in questo modo, con il CIO che fa dei rilievi sulla nuova organizzazione del CONI nel nostro Paese. Quei rilievi sono stati portati all'attenzione del ministro Spadafora; qui ci sono tutti i Gruppi che, insieme al Gruppo del Partito Democratico, hanno partecipato nei mesi passati

fondo. Dispiace che, proprio nel momento in cui si ha il timore di non poter vedere la bandiera italiana, il tricolore, sventolare alle Olimpiadi in Giappone

dispiace perché noi - lo ribadisco - riteniamo che il mondo dello sport abbia dignità e debba essere considerato

che si possa occupare di questo meraviglioso mondo. È un punto al quale teniamo tantissimo. Sappiamo quanto nel Paese vi sia un tessuto connettivo organizzato in associazioni, associazionismo benemerito direi: lo sport di base, gli avviamenti allo sport, le associazioni dilettantistiche, che fanno sì che milioni di persone possano avere in Italia accesso a questo mondo importante, non soltanto dal punto di vista sportivo prettamente inteso, ma anche per tutto ciò che si accompagna alle discipline sportive

che per il resto dell'anno non avevamo considerato e che ogni quattro anni, invece, vengono alla ribalta. Il nostro mondo sportivo è capace di produrre e di lavorare con i bambini e le bambine fin da piccoli per crescere campioni, non soltanto nello sport,

che, insieme agli altri enti pubblici o privati, deve e può fare in modo che tutta l'attività sportiva nel nostro Paese continui a essere quella meravigliosa onda

La politica si deve occupare di sport. Come ho già detto, il Partito Democratico lo ribadisce da sempre. Noi abbiamo votato contro la riforma Giorgetti, che adesso in qualche modo modifichiamo.

nella scuola, con i giovani, interviene nelle situazioni di disagio sociale ed economico. È un elemento importantissimo di sviluppo e di crescita per ciascuno di noi. Lo sport è fondamentale, come già detto, nello sviluppo sociale, a qualsiasi età e in qualsiasi parte del nostro Paese.

tante patologie che possono colpire anche i ragazzi e le ragazze in età adolescenziale, ma ancor di più le persone avanti negli anni.

il tema dello sport, con tutto quanto si porta dietro, debba essere affrontato in maniera completa, esaustiva e approfondita. Ribadisco ancora una volta che per fare tutto questo noi riteniamo davvero che, nel minor tempo possibile, il presidente Draghi debba dare una delega in materia o istituire un Ministero dello sport che se ne occupi.

esame si è reso necessario per ripristinare l'indipendenza del CONI in conformità ai principi sanciti dalla Carta olimpica, soprattutto sulla *governance* e sui finanziamenti. Come è noto, l'Italia ha rischiato di essere sospesa dalle competizioni sportive con l'umiliazione di partecipare senza bandiera e senza l'inno; si era creato un contrasto con la Carta olimpica, che vieta categoricamente a un comitato olimpico di operare per il tramite del Governo e oggi la società Sport e salute

specificatamente individuati. Inutile dire che in sede di discussione in Commissione del disegno di legge delega il nostro Gruppo aveva segnalato le criticità aveva chiesto di attenzionare alcuni passaggi che poi si sono rilevati fatali per le contestazioni del CIO che hanno imposto al Governo una precipitosa marcia indietro. Ci troviamo di fronte al solito caso di una politica che lascia il suo compito di indirizzo, di finanziamento e di verifica dei risultati e si trasforma in un vero e proprio gestore con potere di condizionamento. Non è questo che serve allo sport; non è questo che serviva nella fattispecie. Eravamo stati facili profeti quando avevamo ammonito l'allora maggioranza che si stava percorrendo una strada sbagliata. Noi abbiamo cercato,

Avevamo proposto l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 2, in quanto dall'esame delle tabelle avevamo verificato che con questo tipo di intervento il CONI ha un risparmio di spesa e quindi non c'era bisogno di aggravare il suo bilancio; avevamo proposto un emendamento che ripristinava l'equilibrio tra CONI e Sport e salute spa. Proponevamo, in linea con la legge n. 145 del 2018, una distribuzione di ruoli: Sport e salute SpA ripartisce i fondi e lo Stato vigila sul loro utilizzo. Suggerivamo l'introduzione della temporaneità delle cariche di vertice, per favorire il rinnovamento e anche l'avvicendamento, perché, se non si interviene in questo senso, Riportavamo nella disponibilità di Sport e salute SpA le unità immobiliari destinate all'Istituto di medicina sportiva, in quanto collocate all'interno del complesso Giulio Onesti, *asset* fondamentale per la predetta società, e trasferivamo le proprietà di questo istituto a Sport e salute SpA. Infine, stabilivamo l'autonomia dell'Organizzazione nazionale antidoping (NADO), quale diramazione nazionale dell'Autorità mondiale antidoping. Non è stato possibile discutere questi emendamenti qui vengo anche ad una critica sollevata dal collega del Gruppo Fratelli d'Italia, che vede nella questione di fiducia una sorta di continuità con i Governi precedenti. Ritengo invece che l'odierna posizione della questione di fiducia rappresenti proprio un elemento di discontinuità con il Governo precedente e abbia una finalità di azzeramento. Mi spiego: quello in esame è un provvedimento che non è nato

chiudere la partita, cercando di azzerare il pregresso, insieme a qualche altro provvedimento ancora residuale, in modo che si potesse partire con il nuovo programma e con le nuove iniziative legislative del Governo.

per risolvere le problematiche drammatiche che l'epidemia da Covid-19 ha creato nel nostro Paese. Si tratta infatti di una situazione drammatica dal punto di vista sanitario e dal punto di vista economico, con oltre 100.000 vittime e decine di migliaia di imprese che rischiano il collasso e lo Stato, anche con la proroga della cassa integrazione, ha cercato di mantenere un minimo di livello occupazionale. Vogliamo dunque azzerare e chiudere con il passato,

elemento straordinario e non invece uno strumento ordinario, come è stato fino a poco tempo fa. Quindi, anche se il provvedimento in esame non rispecchia esattamente la nostra prospettiva e la nostra filosofia in tema di sport, assumendoci la responsabilità del momento e anche capendo la finalità del provvedimento - meglio tardi che mai, per ripristinare l'autorevolezza all'interno del contesto internazionale del nostro Paese - voteremo a favore.

meglio tardi che mai: l'Italia ritorna nuovamente a svolgere il ruolo che le compete anche nel contesto internazionale sportivo. Ci auguriamo che in futuro si possa intervenire per migliorare quelle parti e quegli aspetti che non è stato possibile approfondire in questa sede.

Matteoli. Stiamo discutendo di un provvedimento che prevede la possibilità di votare diversi emendamenti. Gli emendamenti sono stati presentati da esponenti del Governo in direzione completamente opposta. La senatrice Sbrollini ha presentato degli emendamenti che considero migliorativi; altri emendamenti sono stati presentati, stranamente identici, da Forza Italia e dal MoVimento 5 Stelle. Poiché questa maggioranza compatta di unità nazionale non ha saputo dirimere la differenza tra questi emendamenti (ecco che «piuttosto che niente, meglio piuttosto»), cosa ha deciso di fare? Ha deciso

A questo punto sono veramente orgoglioso della decisione di Fratelli d'Italia di non partecipare a questo Governo, perché questa è la prima occasione in cui c'è da discutere una decisione presa dal precedente Esecutivo, verso il quale - si immagina - questo Governo voglia mostrare una certa discontinuità

da rispettare, decide di non decidere. Mette la fiducia e lascia tutto impregiudicato, per evitare spaccature all'interno di quella maggioranza che per questo motivo noi non abbiamo voluto supportare. Mai decisione fu più saggia e lo si vede in questo momento. Non è che stiamo parlando di cosette da niente; abbiamo rischiato, a torto o a ragione, che gli atleti italiani alle prossime Olimpiadi partecipassero - pensate - senza la bandiera italiana; quindi non in rappresentanza dell'Italia, ma di se stessi. A questo si è posto rimedio all'ultimo secondo, ma è stata messa una pezza, che rende ancora più colorata la differenza con il resto dell'impalcatura e che oggi viene confermata dalla decisione di apporre la fiducia. Presidente, quando ci spiegano che il contrasto è antico, che il contrasto è tra il CONI e una forza politica che era in maggioranza prima ed è in maggioranza ora, noi che siamo vecchi della politica comprendiamo tutto. Non comprendiamo però l'incapacità di dirimere le questioni politiche. Un Governo che si rispetti, una maggioranza che si rispetti, almeno sui temi che riguardano la rappresentanza dello sport italiano nei confronti del mondo delle Olimpiadi, devono trovare una sintesi;

allora vuol dire che tutte le parole spese sulla possibilità di questo Governo di fare gli interessi nazionali e di trovare soluzioni sono buttate al vento. senatrice Sbrollini ha presentato degli emendamenti; giustamente, secondo me (ma la si può pensare anche nel modo opposto), dice che vorrebbe più fondi e vorrebbe migliorare il rapporto con il CONI e con il mondo dello sport: le rispondono in segno opposto. Non voglio neanche dire

Draghi, che avrà però altri problemi da affrontare. Penso alla pandemia, ai vaccini che non arrivano, ai vaccini che ci sono ma che non sono ancora utilizzati appieno, neanche quei pochi che ci sono; penso penso a quante dosi abbiamo potuto iniettare agli italiani: 1,7 milioni, cioè al 3

anche se è vero che l'Europa in questa vicenda ha fatto veramente schifo (uso una parola poco elegante perché è la verità). Possibile che il Regno Unito, dopo la Brexit, abbia risultati dieci volte migliori? Possibile che gli Stati Uniti d'America, del duo - in questo caso nella stessa direzione - Trump-Biden, abbiano risultati splendidi? Pensate Pensate che negli Stati Uniti, in sette Stati, hanno ormai tolto l'uso della mascherina. Pensate che Israele ha un risultato enorme. Questi sono i problemi che Draghi deve affrontare e io confido che li possa affrontare bene. Fratelli d'Italia è pronta a dargli una mano, se individueremo un piano di vaccini serio e se avremo i vaccini; ma meno male che non ce li hanno dati, che non riusciamo a utilizzare le poche dosi che abbiamo, a chi avremmo dato la colpa se fossero arrivati tutti quelli che erano previsti? Speriamo di risolvere, ma certo, con questi chiari di luna, non si riesce neanche a superare la differenza tra gli emendamenti della senatrice Sbrollini e quelli del MoVimento 5 Stelle e Forza Italia, uniti come un sol uomo (caso più unico che raro,

a trovare una soluzione migliore del voto di fiducia, che fa sì che non cambi niente e rimanga a galla solo una unità di facciata, mentre all'interno il Partito Democratico si frantuma, ma ci siamo abituati. Siamo all'ottavo segretario in pochi anni, cambiano i segretari... *(Richiami

ma almeno risolvete il problema dello sport. Il nostro voto sarà contrario non al provvedimento, ma alla fiducia che il Governo ancora una volta ha chiesto.

con lo sport e che è avvenuto nella mia città, Pordenone, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, dove una giovane pallavolista, schiacciatrice di Carpi - consentitemi il tentativo, improprio in questa vicenda che ha un aspetto drammatico, di rendere un po' più

questo pare l'oggetto del contendere - i diritti legati ad un periodo di attività che ha svolto. Noi sappiamo che il mondo della pallavolo femminile

però non posso non sottolineare che questa vicenda ha suscitato grande attenzione e soprattutto credo non si possa dire che Lara Lugli ha arrecato un danno alla società

che hanno diritto ad avere una vita e non possono essere degli automi. Mi viene in mente il caso delle atlete dell'Est. Non possiamo pensare che il nostro sport diventi di questo tipo, perché veramente vorrebbe dire che la società non progredisce ma torna indietro.

tutti abbiano messo l'accento sulle politiche di genere; il mondo è fatto di uomini e di donne con pari diritti, non è mai superfluo sottolinearlo.

tutelate come dovrebbero, e questo succede perché, se una donna rimane incinta, ovviamente non può avere l'idoneità sportiva a praticare lo sport agonistico, quindi diventa difficile proprio praticare lo sport, ragion per cui bisognerebbe impegnarci tutti a inserire vere tutele a favore delle donne che praticano sport a livelli massimi di agonismo, quindi di professionismo. *(Applausi)*.

provvedimento tecnico e funzionale al completamento di quell'*iter* iniziato con la legge di bilancio di fine 2018, quando la Lega era al Governo. all'articolo 1, commi 629 e 633, si andava a modificare l'assetto organizzativo e il meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva. In quegli stessi commi si attribuiva alla società Sport e Salute SpA il compito di finanziare federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e di corpi civili dello Stato; funzione, questa, attribuita in precedenza al CONI, mentre a quest'ultimo rimaneva il compito di finanziare le spese relative al proprio funzionamento, alle proprie attività istituzionali e alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e a tutto quello che ne consegue. all'esame interviene per ribadire l'autonomia del CONI, così come richiesto dalla Carta olimpica all'articolo 27, che, tra le missioni e il ruolo dei comitati olimpici nazionali, prevede la possibilità per questi ultimi di collaborare con enti governativi e con organizzazioni non governative, ferma restando l'esigenza di preservare la loro autonomia e di resistere a tutte le pressioni politiche, legali, religiose o economiche che potrebbero impedire loro di rispettare la Carta olimpica stessa. Con questo provvedimento il CONI rimane finanziariamente autonomo, con una propria dotazione personale. Quindi, lascerei da parte i tecnicismi e verrei alla sostanza. il nome Sport e Salute promette bene. Fondamentale è stato il passo di distinguere chiaramente quella che è l'attività del Comitato olimpico che si deve occupare di sport in senso stretto, della preparazione relativa alle discipline olimpiche, di tutto ciò che riguarda la promozione dell'attività sportiva e nello specifico dell'attività sportiva competitiva

tempo, purtroppo, si è parlato di sport in modo riduttivo, generico, comprendendo in questa enorme categoria anche tutte le scienze motorie, con le loro figure professionali qualificate, tra le quali, ad esempio, i laureati in scienze motorie. Lo dice una persona che ha vissuto lo sport a tutti i livelli, partendo dallo sport vissuto come attività ludica, sociale e di salute, fino ad arrivare, come dicevo prima, ai massimi livelli del ciclismo femminile. Ho vissuto in seguito lo sport come mantenimento della forma fisica che aiuta il corpo e la mente e infine, purtroppo, l'inattività a cui sono stata costretta ultimamente, che mi dà segnali altrettanto forti di quanto sia fondamentale l'attività motoria per l'equilibrio psicofisico. Purtroppo, in questo anno di crisi sanitaria, economica e sociale, le attività legate allo sport, come tante altre, hanno subito chiusure, sono state sottoposte a regole talvolta senza senso, si sono vietate pratiche di assoluta necessità e si sono consentite pratiche evidentemente in contrasto con la logica. Diciamo che la strada percorsa è stata opposta a quella auspicabile: la prevenzione e la cura preventiva sono state del tutto trascurate. È noto, infatti, come l'attività fisica, specialmente se coadiuvata da figure professionali qualificate, abbia una dimostrata efficacia nell'aumento delle difese immunitarie, mentre su prevenzione, ma anche su cure a casa, siamo stati del tutto inadeguati e deficitari. I giovani sono rimasti esclusi dalle pratiche sportive a seconda del tipo sport praticato o a seconda dell'ente a cui hanno aderito. Non dimentichiamoci che l'agonismo di rilievo nazionale è consentito, quindi molti hanno giocato su questo. Ai giovani è mancata l'attività fisica, la socialità dello sport e il suo insegnamento. Gli anziani hanno avuto danni enormi dal non poter più praticare magari anche quel poco di esercizio fisico o attività motoria finalizzati al contenimento della patologia,

La disabilità, che tanto trova giovamento terapeutico dall'attività motoria, è stata in quest'anno abbandonata al proprio destino. Per non parlare della disabilità mentale, per cui la mancanza di attività fisica ha portato a peggioramenti psicofisici Ebbene, al netto dell'aggravamento della situazione sanitaria evidenziata dal Comitato tecnico-scientifico in questi giorni, l'evidenza è che è a rischio la tenuta psicologica di una popolazione. Attraverso questa azienda pubblica dal nome promettente come Sport e salute auspico prenda davvero inizio una riforma sanitaria in cui la prevenzione sia centrale e l'attività motoria venga posta al centro della questione sanitaria. sanitaria. Quando avremo davvero messo a fuoco questo importante punto, avremo davvero messo in atto un salto culturale a favore del benessere psicofisico degli italiani. *(Applausi)*.

Da sempre noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo battuti e ci battiamo affinché lo sport italiano possa avere un forte rilancio incentrato sulla trasparenza, il riconoscimento della centralità della pratica sportiva non solo come strumento di benessere psicofisico, ma come fondamento di inclusione e aggregazione. profusi molti sforzi e molte misure sono state incentrate sul sostegno al mondo dello sport a tutti i livelli, con il *bonus* ai lavoratori sportivi, i contributi a fondo perduto per centri sportivi, associazioni e società sportive. Un investimento superiore a due miliardi euro per consentire a queste realtà di superare i difficili mesi di chiusura, pur nella consapevolezza che i danni effettivi sono irreparabili. Quello in discussione oggi è uno dei decreti in tema di sport licenziati dai due Governi Conte caratterizzati da importanti novità che hanno avuto il pregio di avviare un cambiamento sostanziale all'interno del mondo sportivo italiano, mettendo al centro delle politiche la promozione e il sostegno allo sport di base, non solo per oggi, ma per i prossimi decenni, favorendo un sano rinnovamento in un mondo che per troppi anni è stato vittima di logiche clientelari. Rilevanti sono il riconoscimento per chi opera nel mondo dello sport e le maggiori tutele per tutti i lavoratori, indifferentemente se a livello dilettantistico o professionistico, ma soprattutto riconoscendo parità e medesimo trattamento alle atlete donne. Per questo motivo la vicenda che ha riguardato un'atleta donna è senza giustificazione, in violazione delle tutele espressamente previste dall'articolo 37 della Costituzione e che le nostre madri costituenti con lungimiranza avevano inserito in questo articolo. Lo sport serve la società, fornendo momenti di eccellenza; ora è giunto il momento di mettere al centro in questo Paese il ruolo sociale rivestito dalla pratica sportiva perché al centro di un Paese in salute risiede la cultura sportiva, valore fondante di una società. Bisogna riconoscere come anche alle persone con disabilità è stata data la possibilità di accedere ai corpi civili e militari dello sport per esercitare l'attività sportiva. In questo senso mi auguro che possa essere approvato il disegno di legge sull'attività motoria nelle scuole primarie, specificando che proprio la sottoscritta ha presentato un disegno di legge in tal senso, che prevede non soltanto l'esercizio dell'attività motoria sin dall'infanzia, ma soprattutto l'insegnamento di una disciplina sportiva - calcio, pallavolo, basket - che possa dare la possibilità a tutti indistintamente, anche ai ragazzi meno abbienti, di avvicinarsi allo sport, interiorizzando le regole e allontanandosi da circuiti devianti, affrontando le tematiche dell'alimentazione e combattendo l'obesità. Come accade nella maggior parte dell'Europa, lo sport è percepito come diritto di ogni cittadino che le istituzioni garantiscono promuovendo un'offerta qualificata e completa che induce ad ampliare sempre di più la base dei praticanti; purtroppo però in Italia non sempre è stato così. Lo sport favorisce l'integrazione anche nei confronti dei soggetti più svantaggiati, per cui sono degni di rilevanza quei protocolli stipulati dal Ministero della giustizia con il CONI o con Sport e salute SpA a favore dei detenuti, adulti e minori. In questo senso occorre sempre più dare la possibilità che queste iniziative possano essere formalizzate. Si chiude oggi un complesso momento riguardante la *governance* del mondo dello sport e l'autonomia del CONI, avendo stabilito una pianta organica per il Comitato olimpico nazionale italiano e l'assegnazione degli *asset* fondamentali per la preparazione olimpica. al nostro esame si è evitato che gli sforzi e i sacrifici dei nostri atleti potessero essere offuscati da una partecipazione alle Olimpiadi senza i nostri colori, la nostra bandiera. Al contempo si è stabilito anche un principio essenziale in base al quale il CONI non potrà muoversi fuori dai paletti di un ente pubblico. Nello specifico vengono assicurate la piena operatività del Comitato olimpico nazionale italiano e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, attribuendo al CONI una propria dotazione organica di personale, anche dirigenziale. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, il testo prevede il trasferimento a quest'ultimo di impianti sportivi e fabbricati specificatamente individuati. Vi è una necessità avvertita da più parti, non più procrastinabile, di una nuova visione che sia in grado di esaltare l'essenza della pratica sportiva dando attenzione alla formazione, all'educazione e alle piccole e medie federazioni; più equilibrio tra promozione e competizione, meno verticismo nella strutturazione del sistema in favore di un modello più inclusivo e partecipato, più investimenti in cultura sportiva dedicando risorse alle istituzioni scolastiche e alle infrastrutture sportive, dovendo segnalare che a tutt'oggi ci sono ancora scuole prive di palestre idonee. A distanza di due anni, che hanno visto due cambi di Governo e l'esplosione di una terribile pandemia, è il momento per tutti di evitare inutili particolarismi, sterili propagande e di cercare, al contrario, un punto di equilibrio sulle norme che possano dare rassicurazione e certezza al mondo dello sport, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità economica del sistema, consentendogli di compiere quel passo in avanti tanto atteso. L'importante nella vita non è la vittoria, ma lottare; la cosa essenziale non è conquistare, ma combattere. Prendendo spunto dalle parole di Pierre de Coubertin, considerato il padre dei Giochi olimpici moderni, ritengo necessario affermare con maggiore forza che il nostro contributo sarà sempre al massimo per cercare le soluzioni migliori. Combatteremo sempre per offrire le soluzioni che la società civile chiede, che il mondo sportivo necessita e che il nostro Paese merita.

dell'articolo unico del disegno di legge n. 2077, di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, nel testo presentato dal Governo al Senato per la conversione.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, che avranno inizio alle ore 13, dopo la sanificazione dell'Aula. Seguirà quindi la chiama, che si concluderà orientativamente

Signor Presidente, con il provvedimento in esame si punta a ricucire la frattura che si è venuta a creare, negli ultimi tre anni, con l'organo di autogoverno del mondo sportivo. Da parte dei due Governi precedenti c'è stato un tentativo di riformare il mondo dello sport. Si tratta di tentativi legittimi, che avevano la loro ragion d'essere nell'importanza che questo settore ricopre per l'economia, per le difficoltà in cui versano molte federazioni, ma anche per alcune cattive *performance* sportive: si pensi alla mancata qualificazione dell'Italia negli ultimi mondiali di calcio. Che però, per via del Covid, ci sia stata una difficoltà di tenuta del sistema è sotto gli occhi di tutti e questo vale per i dilettanti e per i professionisti, per le piccole e per le grandi società, per i gestori e per i proprietari degli impianti, a cominciare da quelli di montagna. Tutto questo rende ancora più urgente una riflessione di sistema sullo sport, attraverso una riforma che naturalmente non intacchi l'indiscutibile principio di autonomia del mondo sportivo e dei suoi organi di governo. Com'è stato stabilito con la risoluzione delle Nazioni Unite del 2014, lo sport, attraverso il Comitato olimpico internazionale (CIO) e le sue filiazioni nazionali, deve godere di massima autonomia per promuovere in ogni parte del mondo i valori dell'istruzione, della salute, dello sviluppo e della pace. Qualsiasi forma di discriminazione è incompatibile con l'appartenenza al movimento olimpico e per sviluppare questi valori universali ne deve essere garantita la massima autonomia e neutralità. Fatti salvi questi princìpi, il mio augurio è che il provvedimento al nostro esame faciliti questa discussione. La pandemia, nelle sue varie sfaccettature, ci ha riproposto tutta l'importanza dello sport. Sentiamo la mancanza degli spettatori negli stadi e, quindi, il valore sociale e di intrattenimento dello sport professionistico. Abbiamo avvertito la mancanza di grandi eventi, come gli Europei di calcio o le Olimpiadi, come fenomeno di festa e di fratellanza fra milioni e milioni di persone. Abbiamo compreso anche l'importanza dello sport di base come strumento per rafforzare le forme di prevenzione primaria, per una popolazione più sana e con sistemi immunitari più efficaci. Oggi l'Italia è un Paese dove tante persone svolgono ordinariamente attività sportiva, ma anche dove ci sono molte malattie collegate a stili di vita sbagliati, come la cattiva cultura dell'alimentazione, che porta il 46 per cento degli italiani a essere sovrappeso. poi dell'obesità infantile, che è tra le più alte d'Europa e rappresenta un'ipoteca negativa sulle condizioni di salute nell'intero arco di vita. Credo che nelle politiche per lo sport la grande questione dei prossimi anni sarà come incentivare una pratica sportiva di massa come elemento ordinario della quotidianità di tutte le persone in ogni fase della vita e, naturalmente, come fare in modo che il movimento professionistico continui a essere una leva della nostra economia e uno strumento di promozione dell'Italia nel mondo. precedente Governo aveva ritenuto di creare un Dicastero specifico per lo sport, dimostrando così un'attenzione particolare a questo settore così importante per il benessere e la salute dei nostri concittadini. Speriamo vivamente

Signor Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, ancora una volta ci troviamo a votare una fiducia al Governo su un provvedimento che proviene dall'Esecutivo Conte-*bis*: un decreto-legge che si è reso necessario per consentire ai nostri atleti di portare alta la bandiera alle prossime Olimpiadi e per far sì che, auspicabilmente, dal gradino più alto del podio possa risuonare il nostro inno nazionale, viste le eccellenze che abbiamo in Italia nel mondo dello sport. È evidente - lo anticipo fin d'ora - che il voto del Gruppo Europeisti sarà favorevole al provvedimento, perché nessuno può assumersi la responsabilità di lasciare i nostri atleti senza il calore di una bandiera e di una Nazione alle loro spalle. Tuttavia, in questa sede mi preme nuovamente sottolineare che, anche su un provvedimento apparentemente semplice come quello in esame, il Governo oggi è stato costretto a porre la questione di fiducia per superare quelle divisioni che esistono e che continuano a manifestarsi anche su provvedimenti non di minore importanza, ma sicuramente di minore complessità.

ma si concretizzi anche nell'effettiva univocità delle azioni che possono farci procedere spediti, anche attraverso un lavoro preparatorio che contempli, nei giorni precedenti la discussione dei provvedimenti, sia nelle Commissioni, sia nei tavoli informali, la capacità di trovare quella sintesi che troppo spesso

sottraiamo al Parlamento e ai singoli parlamentari la prerogativa di intervenire attraverso gli emendamenti e di migliorare quindi i testi. Pertanto, unitamente all'annuncio del voto favorevole da parte del Gruppo Europeisti-MAIE-Centro Democratico, lancio nuovamente un invito a tutte le forze che sostengono questo Governo a concentrarsi sui temi che serviranno a farci uscire dal *tunnel* della pandemia: pandemia sanitaria, ma anche economica.

un elemento fondamentale per la loro crescita equilibrata. Speriamo che, al di là di questo voto di fiducia, che consente di procedere speditamente e di nascondere, ancora una volta, le differenze che esistono all'interno della nostra maggioranza, si possa procedere

È molto tempo che lavoriamo su questo decreto-legge nelle Commissioni competenti e, ne approfitto anche per ringraziare il collega senatore Verducci, che è stato relatore

discutere gli emendamenti che da più parti politiche, a cominciare dal mio Gruppo, sono stati portati all'attenzione delle Aule di Commissione.

perché il mondo dello sport - come tutti i mondi vitali economici, sociali e culturali - da più di un anno soffre immensamente

alle persone più fragili, ai disabili, alle persone che hanno patologie croniche, e a come questo abbia inciso nella loro vita. Ribadisco anche da quest'Aula che l'occasione di parlare di questo decreto mi permette di insistere sul tema. Dobbiamo, accanto al dramma che stiamo vivendo, ripensare alla sicurezza di quei luoghi che sappiamo essere sicuri.

che noi sosteniamo convintamente, il nuovo Governo Draghi. Noi pensiamo, che, in sicurezza, questi luoghi, come tanti altri che stanno riaprendo, debbano tornare alla normalità.

che dovevamo, ovviamente, risolvere un problema immediato: permettere all'Italia di partecipare, come tutti gli altri Paesi, in maniera sicura e normale, con il nostro inno e la nostra bandiera, alle Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno a luglio del 2021. Ma pensiamo anche ai tanti altri eventi che si svolgeranno da qui ai prossimi anni. Penso al grande evento di Milano-Cortina

tornando al testo originale, al testo base senza modifiche, non permetterà al CONI di assumere una piena autonomia. E questo non è uno scontro tra personalismi. Abbiamo delle strutture: ci sono Sport e salute S.p.A., il CONI, e sicuramente altre strutture, che vanno riviste, anche in assenza di un Ministero dello sport, le quali però non devono entrare in conflitto fra loro; loro; strutture che devono svolgere un lavoro preziosissimo, soprattutto per i nostri territori e per lo sport di base, in piena autonomia.

ho evidenziato le ritroveremo a breve e il Governo dovrà mettervi mano, così come dovrà mettere mano, immediatamente, alla riforma dello sport. Ci saranno decreti attuativi sui quali bisognerà porre molta attenzione. Si parla di professionismo femminile, di lavoro sportivo, di tutto ciò che investe anche la quotidianità delle famiglie,

con tanti atleti. Abbiamo fatto un appello - anche sui giornali - oggi in Senato ricordando la vicenda della pallavolista Lara Lugli: addirittura la società ha definito la sua gravidanza

potenziato. E il ministro Elena Bonetti ne ha parlato lungamente anche questa mattina in un'intervista sulla «Gazzetta dello Sport». Bene: credo che, anche su questo, donne e uomini del Senato potranno fare squadra. Pensiamoci bene perché il piccolo passaggio che oggi facciamo dovrà ritornare presto sui banchi del Governo per essere profondamente modificato, e so che anche il Presidente è molto sensibile all'argomento.

del Parlamento ragionamenti che possano poi trovare applicazione, rispondenza e interlocuzione: quello che, invece, in questi giorni è mancato. Lo abbiamo visto e sentito in tutte le salse. Tutti i colleghi che ci hanno preceduto - chi più, chi meno - hanno fatto esplicito riferimento a questo vero e proprio vizio di forma - oserei dire - che ha anche grandi conseguenze di carattere politico. allora a dare un contributo in questa direzione. Non è semplice - ripeto - ma dobbiamo farlo, perché lo dobbiamo ai milioni di praticanti, ai tanti operatori del mondo dello sport, al mondo dello sport stesso che si aspettava

si andrà a porre anche eventualmente come piattaforma per svolgere ragionamenti più ampi, che possano portare in una direzione ben più importante, ovvero quella di una riforma complessiva del sistema sportivo che da tanti anni aspettiamo e che - come abbiamo visto nel corso degli ultimi tempi - non è assolutamente andata a buon fine.

permesso. C'era la necessità di andare avanti in una direzione ben precisa, ovvero dare risposte a un sistema. Il tutto, poi, è stato aggravato da un ulteriore elemento: il mancato conferimento del mandato al relatore; una confusione totale, l'impossibilità di potersi esprimere in qualsiasi direzione sugli aspetti sia migliorativi che peggiorativi. Non è esaltante, anzi - come ho detto - è mortificante. Verrebbe voglia di dire "lo sport, questo sconosciuto".

ma soprattutto di tutti noi cittadini italiani. Vorrei, per un attimo, riavvolgere il nastro e fare qualche piccolo passo indietro per cercare di capire qual è stata l'atmosfera, qual è stato il contesto all'interno del quale è stato emanato il provvedimento. Ricordiamo la spasmodica - oserei dire - attenzione mediatica che è stata ad esso rivolta e il tutto nei giorni precedenti la crisi di Governo. Le possibili sanzioni avevano alzato in maniera esponenziale l'attenzione nei confronti dello sport: tutti gli italiani si stavano interessando a questo problema parallelamente ai problemi legati alla crisi del Governo e, il giorno prima della riunione dell'esecutivo CIO, finalmente il nostro Governo è riuscito ad emanare il provvedimento che ha sanato il *vulnus* e ha di fatto restituito

della caduta del Governo Conte in parallelo a quella dell'emanazione del decreto salva CONI: i nostri atleti erano salvi. C'è stata un'attenzione mediatica senza precedenti. Non intendo soffermarmi sulle modalità attraverso le quali il CIO avrebbe potuto sanzionare, né tantomeno intendo soffermarmi sugli aspetti di democraticità del CIO e dei suoi comportamenti. Non è questo il punto, non è questo il momento; ci saranno altri Intendo, però, sottolineare come l'elevatissima sensibilità che si è manifestata in quei giorni poteva essere propedeutica a uno sviluppo del ragionamento relativo alla conversione in legge di questo decreto che andasse in un'altra direzione.

di fatto, tradendo tutte le aspettative dei milioni di praticanti, questo strumento, che poteva essere un volano - come ho detto poco fa - per rimettere in moto dei meccanismi di discussione sull'ordinamento sportivo, non è stato minimamente preso in considerazione come tale: è stato considerato in maniera veramente triste, un punto di arrivo piuttosto che di partenza; un punto d'arrivo peraltro fastidioso, perché - come abbiamo visto - la maggioranza non si è messa d'accordo, non ha trovato

purtroppo in totale mancanza di interlocuzione. Quale significato politico dare a quello che sta accadendo nei confronti di questa materia che tutti quanti noi amiamo, almeno a parole? Non lo so. Spero che il Governo, prima o poi, possa darci una risposta. Noi, come opposizione, non possiamo fare altro che vigilare e cercare di aumentare l'attenzione, cercando però non solo di aumentarla, ma possibilmente anche di risolvere i problemi che ad essa devono corrispondere. Questo aspetto, legato all'interesse di milioni di praticanti e di centinaia di migliaia di operatori - come è stato richiamato benissimo ieri da Giorgia Meloni alla Camera dovrebbe in qualche modo portare a risolvere in maniera più incisiva le dinamiche del mondo dello sport che tutti quanti noi, almeno a parole, amiamo, anche oggi invece registra l'ennesima occasione persa.

Si poteva e si doveva andare in questa direzione, ma non è stato possibile. È diventato invece - come ho detto prima - un punto di arrivo che ha sintetizzato tutte le problematiche dello sport italiano tutte le problematiche dello sport italiano nella seppur importante partecipazione alle Olimpiadi. Lo sport però non può e non deve essere soltanto Olimpiadi. È fondamentale per la nostra Nazione costruire una cultura sportiva diversa,

Come si dice in tutte le salse - sta diventando un tormentone - sia gli operatori del mondo dello sport che noi politici non abbiamo saputo dare concretezza alle seguenti affermazioni: lo sport come sano e corretto stile di vita, lo sport come elevazione degli aspetti infrastrutturali e occupazionali economici anche del Paese; tutta una serie di considerazioni che affermiamo in tutte le salse, ma che di fatto non sono riuscite a trovare una collocazione in termini di efficacia all'interno di questo e altri provvedimenti. Lo sport Lo sport meritava una dignità diversa, e non la mortificazione che abbiamo vissuto oggi, perché lo sport è salute - come diciamo in tutte le salse - e merita rispetto. E noi di Fratelli d'Italia faremo del tutto affinché possa essere riconosciuta allo sport la dignità che merita, ma soprattutto il rispetto che

Signor Presidente, signori del Governo, il tema dello sport è uno dei temi costitutivi della natura umana. Gli antropologi ci dicono che è la sublimazione della caccia e della guerra, qualcosa che in qualche modo incarna la natura della modernità. È chiaro che un tema come questo meriterebbe molto di più di un decreto-legge. Questo però è uno dei pochi casi in cui il carattere di urgenza del decreto-legge è assolutamente evidente a tutti e incontestabile. Oggi tutte le forze politiche hanno riconosciuto la necessità di procedere celermente alla votazione

Con oggi bisogna iniziare un lavoro parlamentare serio e rigoroso sul tema dello sport, che provi a fare sintesi delle posizioni evidentemente diverse che esistono tra le forze politiche in quest'Aula, come hanno tentato di fare diversi Governi precedenti senza riuscire ad arrivare alla conclusione di un processo. È evidente che avere anche una figura al Governo dedicata al tema è un fatto necessario e giusto; necessario per la rilevanza generale del tema, ma anche per poter costruire un processo di sintesi. E oggi il relatore in Commissione ha rinunciato di fatto a poter presentare una relazione perché la possibilità di costruire una sintesi non c'era. Dobbiamo chiarire alcuni punti chiave. Abbiamo un Comitato olimpico nazionale, che è fondamentale e garantisce la presenza dell'Italia nelle competizioni internazionali; dobbiamo rafforzarlo e sostenerlo. Abbiamo una rilevanza dello sport di base in cui noi crediamo in maniera profonda. La storia del Partito Democratico è di forze politiche di forze politiche popolari che hanno investito nella loro tradizione e nelle organizzazioni sportive di base come elemento di crescita democratica. Lo sport è sicuramente un elemento che riguarda la salute fisica delle persone; è sicuramente un luogo che riguarda l'aggregazione e il divertimento, ma è anche uno di quei luoghi dove si impara la pratica delle regole, dello stare insieme tra diversi, il concorrere con l'altro non come nemico, ma come avversario a cui si riconosce - quando è il caso - di essere più bravo e di prevalere. Tale prevalere non è, un sopprimersi, un cancellarsi. È una pratica democratica: si imparano le regole e la democrazia; si impara che in una relazione si sta dentro a un sistema di regole. Tutto ciò oggi è in grande crisi. La pandemia, in questa situazione come in tante altre, ha portato a evidenziare

delle questioni che attraversano la società possono trovare nella pratica sportiva e nell'immagine sportiva degli straordinari messaggi di risposta pensiamo alla lotta al razzismo e alle differenze - oppure completamente sbagliati e contrari. Noi crediamo - in particolare, lo abbiamo sottolineato come Gruppo - che la funzione dello sport femminile, la piena partecipazione e le pari opportunità delle donne nello sport siano degli elementi fondamentali per rendere più equa, paritaria e più uguale nella differenza la nostra società.

investendo sulla pratica sportiva. Per tutte queste ragioni pensiamo che quello di oggi sia un passaggio necessario, dovuto e assolutamente adeguato,

Ci siamo confrontati sul decreto in maniera civile. Sono emersi punti di vista diversi ed è stato accettato anche il voto di fiducia in maniera assolutamente condivisa. È il clima sicuramente di questo Governo, ma in questo caso ha riguardato anche alcune delle forze dell'opposizione. Partiamo da questo punto e facciamone tesoro; facciamolo diventare una priorità parlamentare di quest'Assemblea e chiediamo con forza, nel messaggio conclusivo anche di questa nostra dichiarazione, che ci sia una figura al Governo che possa diventare il nostro riferimento e con cui dalle prossime settimane si possa iniziare a lavorare per dare allo sport italiano tutte quelle risposte di cui c'è bisogno e che oggi ancora non ci sono.

dell'atleta di Pordenone che è stata discriminata solo per il fatto di aver comunicato il suo stato di gravidanza; questo la dice lunga

ciò sia molto importante e significativo, altrimenti è solo *business*, è solo un fattore economico, pur rilevantissimo (non dobbiamo certamente essere ingenui o delle mammole).

che i nostri atleti e le nostre squadre possano concorrere con la bandiera e nel nome del nostro Paese, ma non facciamo ricadere tutta la questione dello sport nell'oblio, soprattutto per quanto riguarda la sua funzione sociale,

oggi va a completare la legge n. 145 del 2018. Si vanno a delineare i confini di azione del CONI e della società Sport e Salute. Finalmente sappiamo chi, cosa e soprattutto come dovranno agire entrambe le strutture. Io penso che, grazie a questo decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, finalmente il CONI implementerà non solo le sue risorse in termini di liquidità (se non sbaglio avrà circa 6 milioni di euro

Allo stesso tempo, la società Sport e Salute finalmente avrà un quadro e una cornice in cui agire; nessuno ha mai messo in discussione né l'autonomia del CONI, né il fatto che entrambe le società potessero divergere, perché svolgono ruoli totalmente diversi. rappresentante del Governo, svolge una funzione legata allo sport di alto profilo e alle grandi competizioni, mentre Sport e Salute - come ha detto bene la collega che mi ha preceduto - si occupa dello sport di base,

ristori. Le due funzioni possono quindi interagire senza intralciarsi l'una con l'altra? Assolutamente sì. La sfida, cari amici - lo dico senza alcun infingimento, perché forse il dibattito dovrebbe uscire un po' da questa cappa è quella di dire che, a differenza di quanto sostenuto da una collega poco fa, non c'è stato uno scontro di potere o per il potere tra il CONI e la società Sport e Salute. È sbagliata questa interpretazione.

su indicazione del presidente del nostro Gruppo, senatrice Bernini. No alle tifoserie e sì ad ogni sforzo per trovare una sintesi tra le posizioni. Questo è stato l'atteggiamento del Gruppo di Forza Italia in Commissione.

Questa è la vera sfida. Oggi in Parlamento, grazie alla saggezza del Presidente della Repubblica, abbiamo avuto la capacità di cancellare, anzi, di accantonare le nostre differenze per convergere su una sintesi che si chiama presidente Draghi, nell'interesse del Paese. Sarebbe sbagliato se questo spirito non venisse colto, non tanto dal mondo dello sport che lo attende, ma da chi lo rappresenta. Questa è la vera sfida che abbiamo dinanzi e - ripeto - non dobbiamo commettere l'errore di essere partigiani o tifosi degli uni o degli altri. Ho conosciuto ho avuto modo di apprezzare il Presidente del CONI, quando ero Presidente di un municipio di Roma. Ne ho apprezzato le qualità di uomo capace di fare inclusione sociale, che ha messo a disposizione del nostro territorio un prestigioso circolo nazionale di cui era Presidente. La stessa cosa possiamo dire anche del dottor Cozzoli, uomo di Stato, uomo delle istituzioni, che ha rinunciato al ruolo di capo di gabinetto per dedicarsi alla sua passione, allo sport. Oggi affrontiamo questo tema e siamo convinti che tutti quanti noi possiamo cogliere questa sfida. È ovvio che la partita non è chiusa; è ovvio che da oggi si può aprire un nuovo tavolo, augurandoci di avere un rappresentante del Governo che dia dignità al mondo dello sport, che francamente se lo merita, e che ha già pagato un prezzo elevatissimo, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto,

sia chiaro, nessuno di noi vuole essere incosciente - però quello dello sport è un mondo che purtroppo paga un prezzo elevato e noi oggi non possiamo fare finta di nulla. Io spero, anche come membro della Commissione bilancio, che a breve finalmente

abbiamo la necessità che il decreto-legge che andiamo a convertire diventi finalmente legge e che si dia finalmente chiarezza nelle competenze e nelle funzioni; nessuno

ringrazio innanzitutto il sottosegretario Bergamini perché, come è già stato detto in altri interventi, si è ritrovata questa patata bollente - mi si consenta il termine

per un caso strano, trova un consenso pressoché unanime perché si tratta di un decreto-legge che doveva essere emesso in quanto emergenziale, cioè in un momento di urgenza

perché anche la senatrice Sbrollini poco fa diceva che con questi numeri non si poteva garantire appieno l'autonomia del CONI.

che è quello di far conoscere lo sport nelle sue qualità migliori, come quella di poter crescere ed educare; molti colleghi hanno richiamato grandi e bei principi che io sottoscrivo perché lo sport serve a combattere le differenze,

che non viene abbastanza sottolineato. Dobbiamo riuscire a creare un vero ambiente propositivo e positivo, perché

lo sport sia degnamente considerato ed uso appositamente questo termine, perché si tratta proprio di dignità. Non ci sono semplicemente coloro che utilizzano le associazioni sportive per mascherare attività commerciali, ma ci sono anche quelle persone - sono la maggioranza

abbattere le differenze, se si riconosce dignità a coloro che lavorano all'interno di questo comparto.

la sua vicenda ci consiglia di continuare a lavorare sullo sport e su tutte le esigenze, oltre a questa specifica che riguarda la legge n. 91 del 1981, connesse al professionismo nel mondo dello sport. Ci spinge a valutare che sono molte le questioni sulle quali dobbiamo intervenire rispetto al mondo dello sport, non ultima, appunto, quella dei ristori che il settore dovrebbe ancora ricevere.

per tutte le numerose questioni che abbiamo la necessità di affrontare nel mondo dello sport. Lo sport per sua natura è il regno dell'azione fisica umana e, come tale, vive della passione e del vigore atletico di chi lo pratica. Dunque, da sempre, per permettere la sussistenza dello sport, si è profilata la necessità ineludibile di sancire un insieme di precetti e regolamenti che ne consentissero un razionale svolgimento, senza senza intaccarne natura ed essenza, coinvolgente il diritto di esplicarsi in maniera tutelata e tutelabile, *erga omnes*. Da qui l'autodichia del mondo dello sport, dalle gerarchie istituzionali più alte, come quelle del CIO a livello internazionale, a quelle dei comitati nazionali, come il CONI, a cui aderiscono le varie federazioni sportive dei singoli sport. questo principio universale, valido in tutto il mondo CIO, era stato messo in pericolo e bersagliato da un insieme di disposizioni di un recente passato, mal calibrate rispetto all'assunto da cui siamo partiti; anzi, dall'assunto su cui si basa lo sport professionistico a livello mondiale. Il *vulnus* era palese ed era necessario intervenire con buon senso e pragmatismo. La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2021 rendeva noto che sin dalle prime interlocuzioni informali, nonché nelle missive indirizzate dal Presidente del CIO al ministro Spadafora, era emerso l'avvio da parte del CIO di un'attività istruttoria per comprendere gli impatti che la legge n. 145 del 2018 aveva avuto sull'assetto organizzativo del CONI e sul principio di autonomia e indipendenza sancito dalla Carta olimpica. Il CIO aveva dunque rappresentato - e diremmo anche giustamente - all'Italia una serie di doglianze sul ruolo, l'ammissione, l'autorità e le responsabilità del CONI, assoggettato al rispetto dei requisiti minimi della Carta olimpica. In particolare - proseguiva la relazione illustrativa - è stato eccepito che il personale del CONI non potesse essere assunto e controllato da un'entità esterna riconducibile allo Stato (quindi Sport e Salute SpA), ma dovesse avere una propria dotazione organica e una struttura amministrativa. Da qui la necessità di porre rimedio dal punto di vista legislativo con il disegno di legge che ci apprestiamo a votare e - mi si consenta - da qui l'incisiva capacità del Governo Conte di operare, seppur *in extremis*, attraverso le disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2021, composto di quattro articoli e due allegati, che mira dunque ad assicurare la piena operatività del CONI, nonché la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, attraverso la ricostituzione della pianta organica e l'assegnazione dei beni strumentali necessari all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto dei principi della Carta olimpica e, in particolare, dell'articolo 27, comma 6, che, come detto, stabilisce l'autonomia e l'indipendenza dei Comitati olimpici nazionali. Ciò soprattutto in vista, come già detto dai colleghi, della partecipazione della delegazione italiana alla 32a edizione dei Giochi olimpici di Tokyo, che ci auguriamo tutti comincino il 23 luglio prossimo. Stiamo parlando, quindi, di una vetrina planetaria, meravigliosa e imponente, dentro la quale non si poteva permettere che la nostra cara Italia, riconosciuta dalla storia come la patria del bello, non si presentasse agghindata dei suoi vestiti migliori, più eleganti, nelle sue forme più lucide e geometricamente ineccepibili. Infatti, colleghe e colleghi, purtroppo - è bene ricordarlo - si era caduti nella tentazione di politicizzare lo sport e a questa avventatezza siamo stati costretti a riparare. La norma che stiamo votando riporta l'autonomia dello sport al centro del villaggio - parafrasando così un linguaggio che in genere viene utilizzato proprio per le Olimpiadi depotenzia il processo di ingerenza politica nella piena operatività del sacro percorso di autodichia sportiva. Notevole è la qualità della disciplina innovativa che si sottopone alla nostra attenzione e alla nostra responsabilità di legislatori. Si dispone che il CONI sia fornito di una propria dotazione organica nella misura massima di 165 unità di personale, delle quali 10 di personale dirigenziale di livello non generale, in modo da poter essere pienamente operativo, autonomo e indipendente, in qualità di componente del Comitato olimpico internazionale. La dotazione organica consente al CONI di espletare i compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali. Si prevede che il personale di Sport e Salute, già dipendente del CONI alla data del 2 luglio 2002, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (30 gennaio 2021) presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, venga trasferito nel ruolo del personale del CONI, con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata in base alla tabella di corrispondenza richiamata al comma 4. Un'ulteriore disposizione stabilisce che, espletata la procedura di trasferimento del personale verso il CONI o di opzione per la permanenza in Sport e Salute, il completamento della pianta organica del CONI avverrà mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. Signor Presidente, per questa serie di ragioni, che correggono anomalie gestionali precedenti e sanciscono la primogenitura autodeterminativa e la preminenza autonomistica dello sport e dei suoi organi di rappresentanza, organizzazione e funzionamento, a nome dell'intero Gruppo MoVimento 5 Stelle dichiaro il voto favorevole su questo provvedimento.

17 febbraio 2021: fiducia bulgara senza un perimetro di area politica al Governo Draghi. Al Senato 101 voti in più rispetto ai 161 necessari: 262 voti a favore. Eppure, tre settimane dopo siamo già alla seconda questione di fiducia. Come mai? È necessario È necessario rivedere le dichiarazioni in Aula di quel giorno difficile. Tutti intenti a recitare il proprio e personale libro dei sogni, evocati, forse, dal nome fiabesco del neo Presidente del Consiglio. Anche un modesto osservatore come può essere la sottoscritta, però, non poteva che vedere in questo una pantomima. Siete stati messi tutti in un'arena dove lo scontro politico, inevitabile, non potrà che portare ad esautorare il Parlamento delle proprie prerogative e portarlo a non operare. Votiamo no alla fiducia che ci viene chiesta per la terza volta in tre settimane. Non sarebbe stato un no al provvedimento, perché è un atto dovuto, ma non sarebbe stato un no se la Commissione e il Senato avessero potuto essere chiamati ad esprimersi su questo e se avessero potuto contribuire a migliorare il provvedimento. In materia di prerogative parlamentari negate, a questo punto non posso esimermi dal denunciare anche il fatto che l'atto ispettivo, a prima firma della senatrice Fattori, che io ho sottoscritto, sulla vicenda che ha interessato la McKinsey, società di consulenza privata cui il Mef ha dato un mandato di collaborazione, è stato fermato in Presidenza, perché tema delicato, all'attenzione del Presidente del Senato. Il Parlamento è stato svuotato e lo dimostra anche il fatto che le Commissioni stanno faticosamente lavorando, da settimane, su un vecchio *recovery plan* che non è più attuale. Ben consci che i tempi, ma soprattutto la volontà, faranno sì che il Parlamento sarà chiamato solo per essere informato dal Governo sul documento

Non come una società internazionale di consulenza strategica manageriale, *leader* nel mondo per quote di mercato.

non tanto per gli assembramenti, che non tocca a me sciogliere, ma per non disturbare il collega Signor Presidente, come è stato evidenziato più volte, ancora una volta questo Governo ha deciso di porre la questione di fiducia, mortificando Il Parlamento. E lo ha fatto per evitare che il Parlamento discutesse e migliorasse un provvedimento sullo sport, che non migliora lo sport, non risolve i problemi dello sport, che trasuda la visione spartitoria di potere e di *business* che questo Governo e questa maggioranza hanno anche nei confronti dello sport. Il decreto aumenta i posti dirigenziali e non fa nulla per evitare che il Presidente del CONI possa ricandidarsi per più di due mandati. Per noi, lo sport è inclusione sociale, è superamento dei propri limiti, è gioia e possibilità di partecipare. per voi, è business e potere. Ma alla vostra visione un'alternativa c'è ed è per questo che noi voteremo no, anche a questa fiducia.

possa vincere lo scudetto. Nel 1970 il Cagliari vinse lo scudetto contro tutti e contro i pronostici, ma ebbe la possibilità di giocare la partita. la partita. Mettendo sempre il voto di fiducia, impedite al Parlamento di giocare la partita. Il rischio è quello di non avere una ricaduta degli emendamenti, alcuni dei quali erano anche positivi, propositivi e migliorativi, ma non date la possibilità di giocare (altro che De Coubertin). Qui siamo ormai alla violenza delle regole. Viene impedito l'equilibrio delle parti in partita, dei ruoli. L'opposizione è quasi soffocata in un ruolo marginale; siamo costretti a intervenire in dissenso, perché ci viene quasi impedito di organizzarci

date la possibilità alle opposizioni di fare opposizione, esattamente come alle palestre di sopravvivere. Non c'è alcun'eco di sopravvivenza verso un mondo sportivo che da un anno continua a pagare affitti

decreto-legge invito il Governo, per piacere, e anche la Presidenza ad avere un po' più di rispetto verso le parti cosiddette deboli, verso le opposizioni. Dateci la possibilità di giocare la partita, basta con questi voti di fiducia.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

Russo

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2077, di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, nel testo presentato dal Governo al Senato per la conversione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

subita da una ragazza di ventidue anni a Villa Giordani fa piangere Roma; perché l'aggressione, subita sempre da una donna, nell'ex Istituto Mafai a Tor Marancia fa piangere Roma. Violenze passate inosservate, ormai semplice cronaca, ma noi della Lega non vogliamo farle passare inosservate. Siamo qui a denunciare il degrado cui versano alcune periferie di Roma. Lo denunciamo con forza. Ci appelliamo al sindaco Raggi, sempre più assente, sempre più protesa alla campagna elettorale che alle priorità dei cittadini, tra le quali Per questo mi appello al nuovo Governo, mi appello al Ministro dell'interno, ma soprattutto al Sottosegretario Molteni, che già

quattro righe su alcuni giornali locali, nessuno ne ha parlato. Noi siamo qui a denunciarlo. Per la Lega la sicurezza è una priorità; non ci abitueremo mai alla violenza, soprattutto nei confronti delle donne, delle persone fragili,

Signor Presidente, è trascorso un anno dall'inizio del primo *lockdown* nazionale; un anno in cui la pandemia ha provocato profondi sconvolgimenti sociali, ha stravolto il vivere comune e soprattutto ha determinato la più importante crisi mondiale, non solo sanitaria, che ad oggi ha causato la perdita dolorosissima, solo nel nostro Paese, di oltre 100.000 vite umane. Nessuno poteva prevedere che, dopo un anno, le complesse problematiche e la profonda crisi globale sarebbero state ancora in atto nelle loro multiformi sfaccettature e nelle loro poliedriche ripercussioni sulla vita della collettività. #Iorestoacasa era lo *slogan*, il messaggio che aleggiava nei nostri cieli e che rappresentava molto più di un semplice invito. Era un motivo di condivisione, di sentirsi compartecipi di una guerra, difficile e dura, da combattere contro un nemico invisibile che non fa sconti a nessuno, capace di scaricare la sua enorme aggressività e patogenicità soprattutto sulle persone più deboli e più fragili, ma al tempo stesso capace di colpire anche i giovani o gli adulti forti e resistenti. un virus che mantiene la sua forza penetrante soprattutto per la capacità di mutare e di trasformarsi in varianti più aggressive e contagiose; un nemico capace di far sentire i suoi deleteri effetti un po' ovunque. La sua estrema aggressività e la sua rapida diffusione sono purtroppo facilitate e alimentate dai nostri comportamenti sbagliati, dal mancato rispetto delle misure di sicurezza individuali e collettive. Quest'anno è trascorso nel combattere in tutti i modi il Coronavirus, provando a trovare il giusto equilibrio tra le necessità sanitarie indifferibili e la salvaguardia della vita umana, da un lato, e le gravissime problematiche sociali ed economiche dall'altro, che hanno falcidiato il nostro tessuto sociale; tutto ciò cercando di calibrare la pesantezza e l'incidenza dei provvedimenti adottati. A un anno di distanza, la situazione generale, purtroppo, è ancora grave nella sua drammaticità e complessività. Solo un raggio di sole sta, poco alla volta, rischiarando questo cielo plumbeo: i vaccini, che la scienza e la ricerca sono riuscite ad allestire in breve tempo. Un'arma potente che, nonostante le difficoltà legate all'approvvigionamento delle dosi, non ancora sufficienti, alle diverse criticità nell'organizzazione, nella distribuzione e nella somministrazione delle stesse, con la presenza di notevoli sperequazioni tra Regione e Regione, rappresenta comunque il punto fermo da cui partire, permettendoci di infliggere un colpo mortale al Covid-19 e ai suoi deleteri effetti. Le varianti del virus impongono senso di responsabilità da parte di tutti e misure adeguate da rispettare con rigore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è vaccinato a un anno dal primo *lockdown*, con compostezza, serenità e rispetto per la grave situazione che stiamo vivendo: un esempio per tutti noi e anche per i pochi indecisi sulla necessità e imprescindibilità di vaccinarsi. Un messaggio di speranza per il nostro Paese e di sacro rispetto per le oltre 100.000 vittime del Covid.

un percorso che questa Nazione deve assolutamente compiere, che non nasce esclusivamente tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma da azioni che questo Parlamento ha già messo in campo. Mi riferisco, ad esempio, ai tentativi che abbiamo fatto per ridurre l'inquinamento dell'aria.

Signor Presidente, nei giorni scorsi è stato firmato un contratto con McKinsey per la riscrittura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che dovrà pianificare l'impiego dei 209 miliardi, ridotti a 191,5 in arrivo dall'Unione europea. Secondo i giornali, sarebbe stato il ministro Franco a contattare la società. I termini del contratto non sono noti, si sa solo che McKinsey dovrebbe ricevere 25.000 euro per lavorare al più importante progetto di politica economica del Dopoguerra; una somma irrisoria, per affidare il contratto senza alcuna gara a evidenza pubblica, tanto che la notizia è trapelata grazie a Radio a Radio Popolare. Il Tesoro ha diffuso una nota in cui precisa di essersi avvalso dell'articolo 36, comma 2 del Codice degli appalti relativo ai contratti sotto soglia, omettendo il comma 1 dello stesso articolo che recita: «L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto degli altri principi (articolo 30, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti), in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese». E McKinsey non può essere definita piccola o media impresa, tantomeno McKinsey è nota per essere stata dietro numerose decisioni discutibili care ai neoliberisti, essendo stata accusata negli Stati Uniti di aver esacerbato le disuguaglianze sociali, collaborato con l'amministrazione Trump nelle politiche repressive contro l'immigrazione; condannata a pagare 472 milioni di dollari per il ruolo nell'epidemia di oppioidi che ha fatto migliaia di morti l'anno per aumentare le vendite del farmaco oppioide Oxycontin, incoraggiando i medici a prescriverlo in dosi sempre più forti anche quando non era necessario; di aver aiutato il regime saudita in un'operazione di *maquillage* mediatico, per individuare opinionisti e dissidenti che pubblicavano su Twitter opinioni sgradite alla corona saudita; accusata di aver creato una squadra di *troll* che perseguitava il giornalista ucciso Nel 2015 il governo Renzi si avvalse delle analisi di McKinsey per approntare la riforma della buona scuola, contestate dai docenti, poiché basate su tesi economicistiche, che contrastavano quelle socio-pedagogiche, che avevano guidato le riforme della scuola nel Paese. Con le università più antiche del mondo, migliaia di docenti e ricercatori pubblici già pagati dallo Stato, che insegnano alle generazioni future come stilare un piano, con un Governo che si fregia di aver messo nei Ministeri chiave tecnici esperti ed il Governo dei migliori, sfugge il ricorso ad una società privata straniera con accesso a informazioni strategiche, e sfugge la *connection* tra i *club* Diplomatia e Canova, frequentati da soci illustri, alti esponenti dello Stato e aziende pubbliche e private come CDP, Open Fiber, Tim, Banca Intesa, Poste, Fincantieri, Atlantia, Allianz e le banche di affari Rothschild e JPMorgan con Federico Ghizzoni e Stefano Balsamo. La ringrazio, signor Presidente, e spero che d'ora in poi tali interrogazioni, falcidiate dalla mannaia della circolare bavaglio, non siano più censurate. *(Applausi)*.

le comunico con piacere che proprio oggi è stata autorizzata la pubblicazione delle sopraddette interrogazioni. *(Applausi)*. Mi rallegro anche che queste forme aggregative abbiano portato, dopo la nascita di nuovi Gruppi e componenti, anche alla nascita della componente degli interventi di fine seduta.